L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea

apre una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito all'unanimità modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 27 giugno. La discussione in Assemblea del decreto-legge sblocca cantieri avrà inizio nel pomeriggio di domani, con seduta dalle ore 15 alle ore 20. Il calendario prevede inoltre sedute senza orario di chiusura giovedì 30 e, se necessario, venerdì 31. Resta confermato il *question time* di giovedì 30, alle ore 15, con la partecipazione dei Ministri dell'interno, della difesa e delle politiche agricole. La prossima settimana saranno discussi i seguenti provvedimenti: disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica concernente la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni; disegno di legge sul contrasto alla circonvenzione degli anziani; ratifica con il Kenya sul Centro spaziale Luigi Broglio; risoluzione della Commissione agricoltura sull'invasione della cimice marmorata asiatica; mozioni sul contrasto ai cambiamenti climatici, nella giornata di mercoledì 5 giugno, in concomitanza della giornata mondiale dell'ambiente; mozioni su Radio Radicale. La discussione delle mozioni sul contrasto ai cambiamenti climatici prevede, per ciascun Gruppo, 10 minuti comprensivi di illustrazione

sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Nella settimana dal 18 al 20 giugno saranno discussi il decreto-legge concernente misure urgenti per il servizio sanitario della Regione Calabria - in corso di esame presso la Camera dei deputati - e, ove conclusi dalle Commissioni, i disegni di legge sul salario minimo orario, sulla videosorveglianza e sul distacco di Comuni dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna. Mercoledì 19 giugno, alle ore 9,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019. I tempi della discussione sono stati ripartiti tra i Gruppi. Nella settimana dal 25 al 27 giugno saranno discussi i seguenti provvedimenti: decreto-legge crescita economica, attualmente all'esame della Camera dei deputati; legge di delegazione europea 2018 e connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ove concluse dalla Commissione; ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri; seconda deliberazione sul disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari; ove conclusi dalle Commissioni, il disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*, approvato dalla Camera dei deputati, e, dalla sede redigente, il disegno di legge sulla tutela delle vittime di violenza di genere. Mercoledì 26 giugno, alle ore 9,30, avrà luogo la chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di due componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Nelle giornate di giovedì 20 e giovedì 27 giugno, alle ore 15, si terrà il *question time*. Infine, in relazione a diverse richieste di deroga indirizzate alla Presidenza dai Presidenti delle Commissioni permanenti, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che, ferme restando le eccezioni già previste per i decreti-legge e per i pareri su atti del Governo di imminente scadenza, nelle settimane dedicate ai lavori dell'Assemblea le Commissioni potranno riunirsi esclusivamente in orari antecedenti l'inizio della prima seduta

cinque giorni fa a Genova oltre 1.000 persone si sono radunate per protestare contro la manifestazione organizzata da CasaPound nel cuore del centro cittadino. Io stesso, avendo il mio ufficio proprio in tale zona, ho potuto vedere di persona i fatti accaduti: una parte dei manifestanti ha tentato di impedire con la violenza il comizio del predetto movimento di estrema destra, attaccando le Forze dell'ordine che presidiavano piazza Marsala. Negli scontri sono rimasti feriti due carabinieri, a cui va la mia solidarietà e il mio augurio di pronta guarigione. Nel censurare le violenze commesse a danno delle Forze dell'ordine e pur tenendo presente la situazione di tensione e pericolo venutasi a creare, devo tuttavia porre l'attenzione sulla reazione immotivatamente violenta che alcuni appartenenti alle Forze di polizia hanno posto in essere nei confronti del giornalista Stefano Origone. Com'è noto, il pestaggio a cui è stato sottoposto il predetto giornalista è oggetto di indagine da parte della procura genovese, la quale tuttavia sta incontrando difficoltà nell'individuazione degli agenti coinvolti nel fatto. Come già avvenuto ai tempi del G8 di Genova del 2001, il casco, la maschera antigas e la divisa rischiano di rendere indistinguibili i pochi agenti che hanno trasceso dai tanti che, con professionalità e dedizione, compiono il proprio dovere dosando la forza anche in frangenti di stress e pericolo. Per tale motivo auspico che anche in Italia, come già in altri 15 Paesi europei, venga finalmente data attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sui codici distintivi delle Forze dell'ordine. Chiedo al Governo di riferire su quali misure intenda introdurre per responsabilizzare e rendere identificabili gli agenti durante i particolari servizi di ordine pubblico e preannuncio il deposito di un'interrogazione in tal senso. *(Applausi

Signor Presidente, alle 10,13 del 21 maggio Barletta è stata epicentro di un terremoto con magnitudo 3,7, profondo 30 chilometri. Data l'energia e la profondità, il terremoto è stato avvertito su una vasta area (circa 2.000 chilometri quadrati), con risentimenti fino al quarto e quinto grado della scala Mercalli, non generando però danni sensibili, ma solo tanta paura. Molto probabilmente si è riattivata una pericolosa struttura sismogenetica (faglia trascorrente destra est-ovest di Barletta). La storia sismica di Barletta non riporta terremoti catastrofici, ma non è per nulla tranquilla. Si evidenziano due forti eventi con epicentri locali, con magnitudo di 5,7 e 5,2, oltre a importanti risentimenti di terremoti vicini. Non è mio scopo spaventare, ma sono convinto che la conoscenza dei rischi sia basilare per evitare catastrofi in seguito a terremoti naturali o a fenomeni del tutto naturali. Dopo il sisma del 21 maggio, nella consapevolezza di un rischio ben maggiore, è opportuno convertire la paura in occasione di riflessione sulla necessità di difenderci dai terremoti. Nel momento del sisma possiamo difenderci con comportamenti idonei, ma per fare ciò occorre un'adeguata educazione al terremoto, esercitazioni frequenti di protezione civile e comunicazioni in tempo reale. Questo sisma, avvenuto in orario scolastico e di apertura degli uffici pubblici, può essere utilizzato come esercitazione reale, per analizzare le operazioni emergenziali attuate e per far sì che, in un possibile terremoto più forte, tutto funzioni al meglio. Ho perciò all'uopo sollecitato il Dipartimento di protezione civile, che ha prontamente accettato, promuovendo un'apposita riunione in prefettura. Tali eventi devono anche essere di sprone per un'azione governativa orientata alla prevenzione. Su tale fronte, purtroppo molto trascurato nel passato, il Governo del cambiamento è molto attivo: dai finanziamenti per la ricostruzione in zone colpite da terremoti alla microzonazione sismica, agli studi di vulnerabilità dell'edilizia scolastica, al sisma *bonus*. Tanto si può ancora fare per mitigare i grandi rischi naturali, a cominciare dalla conoscenza del territorio. A tal proposito, è auspicabile una maggior copertura di stazioni sismiche a mare, studi delle strutture sismogenetiche e dei modelli crostali di velocità di propagazione delle onde sismiche e il completamento della cartografia geologica.

sette anni fa, il 29 maggio 2012, alle ore 9, la seconda scossa per intensità colpì l'Emilia. Fu una scossa di intensità 5,9 della scala Richter, ma risultò più devastante della prima del 20 maggio. Questa scossa colpì le persone mentre erano al lavoro o a scuola; alcuni sono morti per i crolli sul luogo di lavoro. Grande apprensione ci fu tra la popolazione, per il pensiero riguardo all'incolumità dei bambini e dei ragazzi nelle scuole. furono le vittime, sotto i crolli o per malori causati dalle scosse nei diversi giorni dello sciame sismico. Fortunatamente, tutti gli studenti furono tratti in salvo incolumi. Il mio territorio di origine, i Comuni di Novi di Modena, Concordia sulla Secchia, San Possidonio, Mirandola, Medolla, Cavezzo e San Felice sul Panaro a tutt'oggi sono un luogo martoriato. Manca ancora moltissimo per completare la ricostruzione. Soltanto a Novi il 14 per cento delle famiglie, 234 nuclei, è ancora sfollato. Il commissario alla ricostruzione ha preferito privilegiare i Comuni con danni più lievi, che si trovano anche a 60-70 chilometri dagli epicentri, piuttosto che i Comuni più gravemente danneggiati. Così, dopo sette anni, ancora molte persone, nelle situazioni di disagio più grave, si trovano ancora fuori dalle loro abitazioni. Le loro aziende non sono state ricostruite, i luoghi storici delle comunità sono rimasti a tutt'oggi completamente inaccessibili. Vogliamo risposte dalla Regione Emilia-Romagna sulle tante pratiche che sono state ritardate e che non vanno avanti. La spiegazione ricevuta è che quelle complicate vengono accantonate a favore del disbrigo di quelle semplici, una motivazione che non ci soddisfa per nulla, anzi, ci ferisce ancor di più, nel recepire che chi ha più bisogno viene scientemente abbandonato da parte delle istituzioni, mentre chi ha danni più lievi viene favorito. Ancora abbiamo molte questioni su cui interrogarci e chiedere risposte, una di queste riguarda la possibile correlazione tra l'attività sismica nei nostri territori e l'attività di gestione degli idrocarburi nel nostro sottosuolo. Il 17 aprile Peter Styles, Presidente della Commissione ICHESE, avvertiva così la Regione Emilia-Romagna: «Ci sono molti esempi di sismicità indotta generata da attività sugli idrocarburi. Ho scritto in merito 60 pagine di appendice nel rapporto. Ciò è particolarmente vero in regioni come quella appenninica in cui gli impianti di petrolio e gas si trovano in aree sismicamente attive». Il testo era contenuto Il testo era contenuto in una *mail* indirizzata alla Regione e pubblicata da «Report». Nel programma sono stati ripresi elementi inquietanti, quali fughe di notizie, ritardi e pressioni sulla commissione scientifica indipendente, una commissione che già cinque anni fa poneva dubbi ripresi dai quotidiani. Un servizio chiama in causa, tra le altre, la concessione Mirandola, o laboratorio Cavone, ossia l'area che interseca i Comuni di Novi di Modena, Concordia e San Possidonio, nella bassa modenese. Condivido la richiesta del Capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle Andrea Bertani, che ha domandato alla Regione Emilia-Romagna di fare chiarezza. A sette anni dalle scosse sismiche che hanno lacerato l'Emilia, i cittadini meritano risposte, le meritano soprattutto i parenti delle vittime, coloro che come alla Haemotronic hanno visto morire i propri cari sul posto di lavoro e adesso chiedono giustizia allo Stato. Lo Stato deve rispondere al presente appello.

Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, saluto con grande soddisfazione, sicura che molti condividano questo sentimento, l'elezione della dottoressa Marianna Iovanni a sindaco di Venosa, uno dei risultati più incoraggianti delle elezioni comunali di domenica scorsa. Non lo dico solo da orgogliosa portavoce del MoVimento 5 Stelle. La Iovanni, infatti, è da qualche anno una dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali.

È quello l'argomento, Presidente. Come dicevo, la dottoressa Iovanni è da qualche anno una dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali e il suo percorso lavorativo è simile a quello di tanti ottimi professionisti che, invece di trasferirsi all'estero o lasciare il Sud per Regioni che offrono maggiori opportunità, hanno deciso di restare nel proprio territorio e mettere a disposizione della comunità i loro molti talenti, spesso entrando nella pubblica amministrazione dalle porte di servizio, quasi le sole che questa apre loro, per farla brillare della luce che essi stessi emanano. Venosa riparte, grazie alla Iovanni e alla sua Giunta, dal suo straordinario patrimonio culturale, secondo soltanto a quello di Matera, come già dissi qualche mese fa in quest'Aula. Lo fa mettendo il proprio destino nelle mani di una donna che eccelle per qualità intellettuali e per competenza nel settore che oggettivamente dà alla città di Orazio le maggiori opportunità

un'esperienza esemplare da additare a modello a moltissimi borghi del Belpaese. È quasi fisiologico, però, che nello stesso Belpaese ad un passo in avanti ne corrisponda uno indietro. Mi riferisco alla recente selezione per i direttori dei musei statali, avvenuta adottando una procedura ai limiti dell'incostituzionalità, non a caso introdotta dal precedente Esecutivo, che sarebbe stato possibile - oltre che auspicabile - disapplicare. I docenti universitari «di chiara fama», come li vuole il bando, ai quali è stata affidata la selezione, sembrano infatti avere reso concreti i timori della vigilia: che merito e trasparenza, cioè, fossero sacrificati a logiche stantie. Ciò dimostra l'urgenza di superare quello strumento giuridico solo in apparenza corretto, ma troppo facilmente manipolabile *ad libitum*. Confido che i tentativi di interpretazione postuma del bando tesi a giustificare ad ogni costo decisioni della commissione per la Reggia di Caserta, che alla lettura degli atti sembrano essere indifendibili, possa lasciare il posto ad un'onesta riflessione critica. Confido che, partendo proprio dal MIBAC, questo Governo voglia assumersi l'onore e l'onere di fare finalmente del merito e della competenza valori cardine del sistema, allontanando finanche il sospetto di qualsivoglia opacità.